elettronico. (Segue la verifica del numero legale). Colleghi, credo che oggi di votazioni ce ne saranno diverse; quindi eopportuno raggiungere le postazioni e restarci per un certo periodo. Il

fatto molto grave: leggiamo sui giornali che

che il vice ministro Visco ha ricevuto il nuovo Comandante generale della Guardia di finanza. Noi vorremmo sapere se estato fatto un atto formale rispetto alla rinuncia delle deleghe perche´ non capiamo questa azione del vice ministro Visco.

Non ci edato di vedere e sapere se l’accordo all’interno della maggioranza per l’approvazione del testo del decreto e stato raggiunto. Forse, sarebbe il caso di procedere all’inversione dell’ordine del giorno e trattare prima

un articolo esicuramente positivo ed e quello che cancella il vergognoso condono della sicurezza e della tutela della salute sul posto di lavoro.

la sospensione dei controlli per coloro che hanno regolarizzato i lavoratori non elencati nelle scritture dell’azienda.

]da sei mesi in vigore la sospensione dei controlli sulla tutela della salute sul posto di lavoro per le aziende che hanno fatto un condono, che non c’entra nulla con la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.

a mio avviso inquietante, ma – per carita– puo essere una mia preoccupazione. Il vice ministro Visco ha partecipato alla festa della Guardia di finanza. Ha ricevuto il nuovo Comandante generale della Guardia di finanza. Noi sapevamo, perche´ in quest’Aula cosıera stato detto, che erano state ritirate le deleghe al vice ministro Visco. Ora gradirei che la Presidenza

di legge: (1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

che la questione relativa all’adeguamento degli impianti per avere una frazione organica di qualita` venga affrontata all’articolo 9, laddove si parla del nuovo piano e quindi della messa a norma degli impianti.

di 60 giorni almeno uno degli impianti sia in grado di fornire una produzione a norma tale da avere una frazione organica stabilizzata da utilizzare nelle aree individuate nel decreto.

«Cominciata la votazione,» – eil nostro caso – «questa non puo essere interrotta e non epiu concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo

senza contenuti sostanziali, naturalmente, ma solamente a fini propagandistici – aveva evidenziato, ovvero che quei Comuni avrebbero ricevuto,

Adesso il Governo esprime parere favorevole alla soppressione del comma 5 perche´ cosı si leva dagli impacci, come si suol dire, di dover effettivamente attivare procedure che possano portare a compensazioni sostanziali. Noi avevamo invece proposto che tali compensazioni fossero effettivamente

Governo e maggioranza non intendono dare una lira o un centesimo di compensazione a popolazioni alle quali impongono per legge la presenza delle megadiscariche. Credo che sarebbe molto piuserio stabilire che le compensazioni devono essere concesse e stanziare i fondi per erogarle, senza farne solamente un annuncio propagandistico, come era nel decreto originario del Governo, e quindi decidere che cio venga fatto. Questo eun ulteriore segno dell’irresponsabilita del Governo nell’apprestamento del decreto e della maggioranza nel consolidare tale irresponsabilita. il nostro voto sull’emendamento in esame e contrario, perche´ vogliamo che le compensazioni vengano stabilite e vengano definiti in questa sede i fondi opportuni, fuori della tassazione ordinaria sullo smaltimento dei rifiuti, ma a carico dell’emergenza, per le compensazioni a tali Comuni.

raccolta differenziata che auspichiamo venga effettuata anche in Campania.

Presidente, vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi sul fatto che con l’articolo 2, in realta, stiamo disponendo la riapertura selvaggia

partecipazione in Aula e la condivisione di partiti quali i Verdi di Pecoraro Scanio (che tra l’altro e campano) e Rifondazione Comunista, che hanno affermato il contrario per un decennio. per un decennio. Qui oggi prendiamo atto di queste autentiche mostruositaambientaliste ai danni di tutta la Regione Campania. Si tratta di una vera e propria aggressione nei confronti della Regione, perche´ – sia chiaro – nessuno potra dire in Aula di non aver capito che si riapriva una discarica nel Parco nazionale del Vesuvio, che si riaprivano discariche in deroga a specifiche disposizioni in materia sanitaria, ambientale e altro, e, ancora, che si dispone la riapertura di tutti i siti, anche di quelli sequestrati della magistratura. Questo per fare chiarezza.

conseguenzialmente alla scelta dei siti, il tema delle bonifiche e un elemento essenziale che dovrebbe accompagnare in maniera contestuale l’intervento sul territorio. Allora, il senso dell’emendamento se a Bertolaso sono stati concessi ampi poteri, se addirittura con questo decreto si interviene sul rapporto delicatissimo tra poteri dello Stato (e qui poi apriro una breve parentesi), non si capisce per quale motivo

per consentire al commissario delegato di avere un’ampia gamma di possibilitadi trattativa con i territori interessati ed anche per garantire l’intervento di bonifica che finora non e stato mai concretizzato nella Regione Campania. A tal proposito, vorrei dire al senatore Novi che, in realta, lo scenario e ancora piucomplicato.

e giastato attuato con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri perche´ la vicenda di Ariano Irpino si inserisce in tale contesto. In altri termini, il Presidente del Consiglio ha gia utilizzato

Per questo motivo chiedo all’Aula di votare a favore di questo emendamento, al fine di determinare una scelta importante dal punto di vista del sistema e per affrontare correttamente l’emergenza rifiuti in Campania.

Presidente, con questo emendamento non facciamo altro che rispondere alla sollecitazione della Commissione giustizia del Senato che ha giustamente intravisto nel provvedimento del Governo una lesione delle prerogative della magistratura con la possibilita addirittura di utilizzare siti sottoposti a sequestro giudiziario. Riteniamo che l’indicazione data dalla Commissione giustizia del Senato debba essere rispettata sopprimendo, quindi, le parole «anche sottoposti a provvedimento di sequestro» e via via fino alla fine del comma. Cosıfacendo non faremmo altro che dare una risposta positiva alla stessa maggioranza che in sede di parere della Commissione giustizia si e espressa in tal senso. Ma vi edi piu: approvando il precedente emendamento 2.11 della Commissione si eulteriormente allargata la maglia di rapporti anomali tra il commissario all’emergenza e i siti sequestrati, perche´ si e data la possibilitadi passare per strumenti diversi da quello della requisizione, dimenticando che siamo in un regime di emergenza. In un regime di emergenza la requisizione puo anche essere giustificata, ma una trattativa che possa essere tra le parti diversa da quella della requisizione giustificata dall’emergenza diventa assolutamente anomala soprattutto se poi efatta nei confronti di siti sequestrati dalla magistratura. Quindi, per riallineare in termini di costituzionalita questo provvedimento, cosı` come mi ero permesso di sottolineare anche nella pregiudiziale

del senatore Morra ed altri proprio del nostro Gruppo.

senatore Polledri,

dire due cose rapide che riguardano principalmente la questione della discarica di Difesa Grande. Dal piano regionale predisposto dal commissario apprendiamo che i quattro siti dovrebbero essere essere predisposti per l’utilizzo non prima di due mesi e mezzo o tre mesi, stando alle piu rosee previsioni (abbiamo visto peroche in questi sette o otto mesi di gestione di previsione non ne e mai stata rispettata una). C’e` un

mi inchino e sono convinto che verrarispettato, ma la domanda che mi faccio e: cosa succedera` fra venti giorni dato che i primi siti, come dicevo prima, verranno realizzati fra due mesi e mezzo? Credo che il Governo su questo abbia il dovere assoluto di dare una risposta.

tanto premesso: impegna il Governo ad attivare le necessarie iniziative finalizzate a far cessare l’attivita` di stoccaggio di eco-balle nel sito «Taverna del Re», nel comune di Giugliano, entro il 31 ottobre 2007.

all’ordine del giorno G3.101, potrei accedere alla richiesta di modificare il termine entro il quale

come sempre gli ordini del giorno hanno un significato molto preciso di impegno. Ho discusso a lungo con il presentatore, con il Governo e con chiunque abbia preso in considerazione l’ordine del giorno G3.101, che a me francamente appare molto chiaro e soprattutto individuabile nell’indicazione di un unico punto di riferimento, che e` la data temporale. Mettere due riferimenti, ossia la data temporale e il collaudo del termovalorizzarore di Acerra, francamente diventa

ci sembrava quasi ovvio che all’interno del provvedimento in esame si facesse riferimento a Parapoti. Pertanto, mi rimetto all’Aula nel senso che la vicenda Parapoti in qualche modo va affrontata o inserendola all’interno del decreto in esame o, se non se lo si ritiene,

ci dobbiamo soffermare un momento: perche´ non sono possibili nuovi siti? Evidentemente si ritiene che quell’area e stata tipizzata per gli effetti della discarica di Difesa Grande come area a

il Governo successivamente – evidentemente non potevamo chiedere tanto in questa fase al relatore – dovrapensare di sopprimere anche la discarica di Savignano Irpino, che dista dalla localita di Difesa Grande soltanto qualche chilometro in linea d’aria. Allora, se ha senso vietare nuovi siti nel Comune di Ariano Irpino, dovrebbe aver senso anche intervenire sull’articolo 1 e proibire l’attivazione della discarica di Savignano Irpino

non e riuscita a mandare sotto il Governo che in ogni votazione, non aveva i numeri nella sua completezza. Quindi, un richiamo lo voglio fare chiaramente! Pero, torno al merito

sia sui siti sia sulla localizzazione, sia sulla realizzazione dei termovalorizzatori siamo ancora purtroppo in alto mare ed il problema Campania e` un problema di tutti. SODANO (RC-SE). Domando

dire al Governo che questo emendamento e questa soluzione che estata individuata dovrebbe far riflettere anche sull’approccio diverso che in quella Regione si deve assumere rispetto al rapporto con le comunita locali. Ciovale soprattutto per il commissario straordinario. Sono bastati alcuni incontri con gli amministratori per far sı che questi, con grande senso di responsabilita, si facessero carico di un sacrificio di ulteriori venti giorni. quando si evita l’utilizzo della forza per far transitare un camion o un mezzo meccanico e sempre una vittoria della politica e penso che su tale aspetto dovremmo riflettere di piu. Per quanto riguarda le sollecitazioni del senatore Morra, vorrei ricordare che il lavoro di miglioramento del decreto che e stato fatto ha sempre guardato al rispetto delle autonomie locali. Le uniche modifiche che sono state apportate riguardano

con una delibera della Giunta provinciale, come abbiamo anche ascoltato in Commissione, per cui non siamo in presenza di un atto centralistico di imperio ma di una presa d’atto della volonta` dell’amministrazione provinciale. Quindi, in quella sede rivolte le attenzioni o anche le sollecitazioni per comprendere i criteri che hanno portato a quella individuazione. Non potevamo certo interferire con una scelta autonoma della Provincia di Avellino. Credo pertanto che oltre

Che noi stabiliamo con legge di chi debbano servirsi i Comuni della Regione per provvedere allo svolgimento del servizio di raccolta differenziata appare veramente una prevaricazione anticostituzionale. Quindi, questo nostro emendamento non fa altro che rispondere ad una sollecitazione della 1ª Commissione, dove mi pare di capire, come in tutte le altre Commissioni e come in quest’Aula, vi sia una maggioranza allineata con il Governo. Se poi in Parlamento per effetto di giochi, nel senso buono del termine, e comunque di accordi tra relatore, Governo e maggioranza, si disattendono anche i pareri che la maggioranza rende in Commissione, naturalmente se ne risponderain sede politica. Ad ogni modo, vi e una una violazione costituzionale lesiva delle facoltadei Comuni di scegliersi coloro che debbono effettuare un servizio, riconosciuto tra i servizi fondamentali dei Comuni, come quello

formale o costituzionale, Presidente, hanno giadato pessima prova di se stessi. Infatti, se i consorzi sul territorio avessero funzionato, la raccolta differenziata sarebbe ai livelli previsti dalla norma e non vi sarebbe bisogno di un’ulteriore pressione di legge per sollecitarla.

nel senso che la sollecitazione della 1ª Commissione mi pare colga un punto importante sull’autonomia gestionale dei Comuni, cosı come pure l’emendamento da lui illustrato fa riferimento ad una questione secondo noi

siano in condizione di assumere il ruolo che intendiamo assegnargli con una legge dello Stato e non vorremmo correre il rischio di finire dalla padella alla brace. In questo senso, un po’ di cautela rispetto alla, in punto

le considerazioni sviluppate del collega D’Alı` per l’altro emendamento, perche´ sono in stretta connessione, atteso il deficit che tutti riconoscono, anche i colleghi della maggioranza, sull’efficienza ed efficacia dell’azione dei consorzi attualmente esistenti nella Regione Campania.

potrasolo proporre «alla Regione di disporre l’accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento». Cio significa che la decisione

Presidente, durante il dibattito su questo provvedimento ho ritenuto di non intervenire, sia in Commissione che in Aula,

Ora perosiamo di fronte ad un emendamento su cui francamente non posso esimermi dal dire qualcosa. Credo che il collega Novi abbia perfettamente ragione. Quando si nomina un commissario nell’emergenza, lo si fa per snellire le procedure, per far sı che tutto si svolga nel modo piuveloce possibile, per arrivare a raggiungere l’obiettivo.

al coinvolgimento del presidente della Giunta regionale (che ad un certo punto ritenne di volersi dimettere, anche con una certa polemica), poi si etornati a nominare i prefetti; ma mai

I consorzi, nei fatti, hanno la vita segnata dall’approvazione della nuova legge regionale, che avendo ridisegnato i territori campani ed essendo passati da 18 consorzi a 6 Ambiti

Molti di questi consorzi sono giacommissariati e la proposta al presidente e dovuta solo al fatto che, essendo i consorzi di istituzione regionale, non vorremmo avviare un contenzioso rispetto a decisioni del commissario. Nessuno ha intenzione di tutelare strutture inefficienti,

Presidente, la materia emolto complicata e il punto centrale e che il decreto-legge prevede che siano i cittadini della Campania a pagare l’imposta supplementare. presentato dalla Commissione, non risolve in alcun modo il problema e voglio che i cittadini della Campania capiscano e sappiano che l’attuale maggioranza li espone ancora una volta ad un rischio gravissimo. Voteremo contro l’emendamento, perche´ e` una presa in giro rispetto al costo delle tariffe.

di quello all’articolo 7, di rassicurare il senatore D’Onofrio che la congruita che qui si chiede impedira` che i cittadini debbano pagare i costi dell’emergenza: dovranno pagare

credo che l’eliminazione della parola «domestiche» non provochi problemi sotto il profilo finanziario; anzi, a quel punto, si riferisce a tutte le utenze, anche a quelle non domestiche. Quindi, si presuppone che paradossalmente sotto il profilo finanziario l’abolizione della parola «domestiche» sia virtuosa.

Senatore Polledri, il mio estato un eccesso di zelo nel richiedere il parere della Commissione bilancio, che puo essere espresso direttamente in Aula in base all’articolo 100 del Regolamento.

La Costituzione prevede che deputati e senatori possano votare secondo la propria volontasenza doverne rispondere. Non c’e da stupirsi per l’astensione di qualcuno.

consorzi che, come e stato riferito e ricordato anche da altri colleghi, afferisce alla Regione che dovrebbe farlo. Pertanto, confermo il parere contrario Mi sembra che la richiesta di accantonamento non abbia portato a nessuna considerazione delle argomentazioni che avevo svolto e che erano state condivise anche da colleghi della maggioranza.

dal senatore Libe´, propone una questione vera e anche condivisibile. Suggerisco e propongo al collega Libe´ di trasformarlo in un ordine del giorno

anche il sindaco di Napoli, limitatamente alla citta di Napoli, faccia parte dei subcommissari. Si tratta della realtaurbana assolutamente piu rilevante di tutta quell’area ed esiste un voto unanime del Consiglio comunale di Napoli affinche´ il suo sindaco, che poi spesso, anche anche dal punto di vista dell’immagine, eil primo interlocutore non solo dei cittadini ma anche dei mass media nella vicenda, debba essere coinvolto non tanto nella responsabilizzazione, quanto nella

Nel prendere atto che la maggioranza econtro i poteri del sindaco di Napoli, onorevole Rosa Russo Iervolino, e che quindi non la difende piu nessuno,

7 si collega anche all’articolo 8, vorrei capire dal Governo – che non sta rispondendo a nessuna delle domande – dove si intendono prendere le risorse per coprire

7, non per il merito (che comunque mi sembra sconvolgente, perche´ in futuro i Comuni campani non applicheranno le ordinarie misure legislative

e lo scioglimento dei Consigli comunali sulla base di una norma che si applica quando vi sono gravi violazioni della Costituzione, dell’ordine pubblico o di legge, quindi situazioni drammatiche che autorizzano l’autorita`

Se continuiamo a lavorare nonostante la seduta alla Camera sia convocata per le ore 12 si crea un precedente antipatico. Le Commissioni non possono lavorare in concomitanza con l’Aula, figuriamoci se puolavorare l’Aula quando e convocata alla Camera una

e nessuno ha sollevato problemi rispetto alla sua conclusione. Colleghi, c’e una serie infinita di precedenti rispetto a questa situazione.

comunque dieci minuti di sospensione, accogliendo le sollecitazioni dei colleghi su questa parte dell’articolo 7 per le norme